*(PdL)*. Signora Presidente, signor Ministro, colleghi, le recenti prospettazioni dell'OCSE confermano per il nostro Paese una ripresa lenta, selettiva, discontinua, il che rende cruciale il tema dell'integrazione tra le politiche passive e le politiche attive del lavoro. Le chiedo dunque, signor Ministro, come il Governo intenda procedere per integrare politiche attive e politiche passive del lavoro, insieme con le Regioni, da un lato, preservando la dimensione della protezione sociale garantita dagli ammortizzatori sociali e, dall'altro, proteggendo e promuovendo la dimensione della formazione come strumento di connessione attiva e propulsiva tra la persona e il lavoro, mercé l'intermediazione del mercato, muovendo anche dalla constatazione che accordi recenti, proprio con le Regioni, hanno dato risultati di grande interesse. Mi riferisco, da una parte, all'accordo per la destinazione di risorse del Fondo sociale europeo da politiche attive a politiche passive, che ha consentito di finanziare quella Cassa integrazione in deroga che è stato uno strumento formidabile di tenuta della coesione sociale e, dall'altra, signor Ministro, alla recente, profonda ed intensa riforma della *machinery* formativa, che con un accordo - insolitamente sottoscritto persino dalla CGIL - ha posto

Signora Presidente, signor Ministro, colleghi, di fronte alla gravissima crisi occupazionale che il Paese sta attraversando e che ormai è ammessa da tutti, anche dal Governo, il Governo stesso ha scelto di non procedere ad una vera riforma degli ammortizzatori sociali e degli strumenti di protezione del reddito e, soprattutto, di garanzia delle prospettive occupazionali di tutti i lavoratori. Viceversa, è stata messa in atto una sorta di modifica amministrativa degli strumenti preesistenti, integrandola con risorse - come veniva ricordato - provenienti dalle Regioni, e si è creato un *continuum* nell'utilizzo dei diversi strumenti tradizionali. Questa scelta lascia aperti alcuni interrogativi di efficacia e in particolare a questi noi le chiediamo, signor Ministro, di rispondere. Una delle innovazioni è la cosiddetta ordinarizzazione della Cassa integrazione straordinaria; tale termine è utilizzato dal professor Mastrapasqua, presidente dell'INPS. quanti lavoratori abbia interessato, quante aziende e per quante essa sia prossima alla scadenza, poiché ha una durata del 50 per cento inferiore a quella precedentemente prevista. Inoltre, quanto agli strumenti in deroga, che dovevano proteggere soprattutto i settori e i lavoratori non coperti, non è dato di sapere, se non da un'ultimissima tabella dell'INPS, quante aziende, quanti lavoratori e quali settori abbiano interessato, con particolare riferimento (questo ci interessa) alle aziende con meno di 15 dipendenti.

Il Governo, per quanto attento ai conti pubblici, ha dovuto stanziare cospicue somme per interventi di sostegno al reddito a beneficio dei lavoratori sospesi dal lavoro a causa delle difficoltà che, d'improvviso, tante imprese hanno dovuto affrontare. Grazie anche all'accordo con le Regioni, si è provveduto al finanziamento per gli ammortizzatori sociali cosiddetti in deroga che - come lei ben sa - sono linfa vitale per la sopravvivenza di tante piccole e medie imprese. Ora sentiamo di una manovra economica rigorosa, fatta di tagli, di tassazioni, di nuovi *ticket*, di pesanti sacrifici per salvare il nostro Paese dal rischio Grecia, come riportato dalle cronache di stampa. Chiediamo dunque di sapere se ci sono ancora risorse disponibili per gli ammortizzatori sociali, in particolare per quelli cosiddetti in deroga, e quali sono le iniziative che si intende porre in essere a tutela dei lavoratori delle piccole e medie imprese.

nei primi mesi del 2010, le ore autorizzate di Cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che straordinaria o in deroga, sono state ben 415,7 milioni contro le 204,8 milioni ore del primo quadrimestre del un incremento nel periodo stesso del 103 per cento. Pertanto, la Cassa integrazione guadagni straordinaria, che è utilizzata solitamente per le crisi di tipo strutturale, sta crescendo più di quella ordinaria. Questo è un segno molto evidente, e noto a tutti, del fatto che la crisi si prolunga, che si sta cronicizzando, che investe sia le grandi imprese come le piccole imprese e le imprese di servizio. Poiché l'economia del Paese non sta ripartendo, ma si sta consolidando, in negativo, una stasi produttiva piuttosto forte, noi chiediamo di conoscere se e come il Governo intenda adoperarsi perché siano assicurate le risorse necessarie

Signora Presidente, colleghi, signor Ministro, se il biennio 2008-2009 è stato difficile per l'economia mondiale e per il sistema economico italiano, il 2010, avviatosi sotto il segno di una ripresa della produzione e degli scambi internazionali, presenta ancora, come si è visto nelle ultime settimane, forti rischi di instabilità. In Italia la caduta del PIL è stata molto accentuata e più forte di quella registrata negli altri Paesi industrializzati: il PIL è tornato ai livelli dell'inizio degli anni 2000 e, per quanto riguarda il mondo del lavoro, l'ISTAT ha reso noto che, nel marzo 2010, il numero di occupati è vicino a quello registrato a fine 2005 e inferiore di oltre 800.000 unità rispetto al marzo 2008. Il tasso di disoccupazione è cresciuto ed è cresciuto il tasso di inattività. I provvedimenti finora adottati, basati principalmente sull'erogazione della Cassa integrazione straordinaria, si sono dimostrati poco efficaci, sia perché non in grado di dare sicurezza a lavoratori ed imprese, sia perché in molti casi hanno finito per creare sperequazioni nel trattamento. In una simile situazione diventa ancor più urgente una riforma attesa da anni, quale quella degli ammortizzatori sociali; il Governo Prodi aveva tracciato le linee guida per una riforma complessiva degli ammortizzatori sociali con la legge n. 247 del 2007, un testo importante che nasceva da un percorso condiviso con tutte le parti sociali. Il Governo Berlusconi, al contrario, si è fin qui impegnato soprattutto a smantellare o, quantomeno, a rinviare *sine die* le disposizioni di quella legge, limitandosi ad annunciare, con una lunga serie di dichiarazioni mirabolanti, riforme degli ammortizzatori sociali, di cui finora tuttavia non c'è traccia. Chiediamo dunque di sapere quale sia la linea concreta, se c'è, che il Governo intende adottare in merito alla riforma della Cassa integrazione.

vorrei innanzitutto ricordare, in particolare alla senatrice Carlino, che su un punto tutti gli osservatori internazionali, dall'OCSE al recente G20 dei Ministri del lavoro, cui ho partecipato, fino all'Unione europea, in atti ufficiali facilmente acquisibili, hanno riconosciuto che l'Italia ha attenuato l'impatto della crisi generale, dei mercati finanziari prima e delle economie reali dopo, attraverso l'impiego di strumenti che sono stati rivolti alla continuità del rapporto di lavoro, anche quando venivano meno le ore lavorate ed entrava in condizioni di difficoltà non solo il lavoratore, ma anche l'impresa che lo doveva remunerare. Abbiamo realizzato un accordo con le parti sociali e con le Regioni, assolutamente importante per governare insieme questa stagione difficile, in modo tale da mantenere viva la base produttiva e occupazionale. Abbiamo usato strumenti, come appunto la Cassa integrazione nelle sue diverse forme e i contratti di solidarietà che sono stati ulteriormente agevolati, cioè dotati di risorse per una protezione del reddito superiore del 20 per cento, in modo da mantenere viva la base produttiva e occupazionale del Paese

nonostante la caduta della domanda e, quindi, della produzione e delle ore lavorate. In questo contesto, sarebbe stato un errore fare la scelta che ci veniva suggerita dall'opposizione. Mi riferisco alla proposta di impiegare le risorse aggiuntive (quegli otto miliardi aggiuntivi risorse dello Stato per due terzi e dalle Regioni, attraverso il Fondo sociale europeo, per un terzo) sull'indennità di disoccupazione, perché questo - come disse il Segretario generale della UIL avrebbe incentivato la rottura del rapporto di lavoro, anziché incentivare la continuità del rapporto di lavoro. Si fa una riforma nel vivo di una condizione straordinaria? In tali circostanze si fa qualcosa di più rispetto ad una strumentazione ordinaria, anche una riforma non avrebbe dato la dimensione della strumentazione che abbiamo adottato. Non potevamo tarare una riforma su una condizione straordinaria, nella quale si dà di più perché si mette a carico del bilancio dello Stato un'ingente quantità di risorse che altrimenti dovrebbero essere garantite dalla base assicurativa, che è la caratteristica positiva del nostro modello di ammortizzatori sociali, che dovremmo mantenere anche nei percorsi di razionalizzazione. Si adottano misure straordinarie, perché le si prolunga per un tempo che, in condizioni ordinarie, sarebbe ritenuto eccessivo. Ma soprattutto, qual è il tema all'ordine del giorno? Da un lato, certamente, c'è l'esigenza di avere risorse per continuare nell'uso di questi strumenti. Ricordo alla senatrice Ghedini che è stato

Non esiste nessun lavoratore per il quale si sia esaurita la Cassa integrazione ordinaria che poi non abbia potuto accedere ad un altro strumento, come la Cassa integrazione straordinaria per crisi o quella in deroga.

- e soprattutto sono in corso i conteggi per verificare se le somme impegnate sono state poi effettivamente spese, perché una cosa è la dimensione dell'autorizzazione all'uso della Cassa integrazione, una cosa è poi l'uso effettivo, perché se un'impresa ha bisogno di quei lavoratori li chiama al lavoro e non si ricorre fortunatamente all'effettivo uso di una cassa, pur autorizzata. Ma qual è il grande tema ora, prima ancora che parlare di riforma? Vorrei ricordare, tra parentesi, che il Governo Prodi ci ha lasciato una delega senza risorse; una delega di riordino, la cui proroga è stata chiesta nel cosiddetto collegato lavoro all'esame del Senato; ma, sia chiaro, si tratta delega di razionalizzazione dell'esistente, senza aggiunta di risorse. Ebbene, oggi noi dobbiamo combinare quanto più possibile la protezione cosiddetta passiva, cioè l'integrazione del reddito di colui che è costretto all'inattività, con la cosiddetta politica attiva, cioè con l'aggiornamento e il rafforzamento delle sue competenze, in modo tale da renderlo quanto prima nuovamente occupabile, ed accompagnarlo e non lasciarlo solo nella ricerca di un'altra occupazione; e qui soccorrono gli accordi di cui ha parlato il senatore Castro.

per dare attuazione alle intese sul modo nuovo di fare formazione e per ridefinire, proseguire l'accordo relativo ai cosiddetti ammortizzatori sociali. Con le nuove amministrazioni regionali dobbiamo fare in modo che politiche attive e passive procedano di pari passo. Per quanto riguarda la formazione, sono tre i criteri unanimemente accettati e proposti dal Governo.

una sperimentazione circa la certificazione dei mestieri e delle competenze che deve avere una persona che, a sua stessa richiesta, può magari essere effettuata dalle associazioni di categoria, per aiutarla nella ricerca di un'altra opportunità di lavoro; infine, formazione non più per materia in ambito scolastico, anche nei confronti di un adulto o di un giovane in transizione dalla scuola al lavoro, ma formazione per compiti, per competenze in situazione lavorativa. Concludo con una considerazione riferita alle piccole imprese, alle imprese con meno di 15 dipendenti,

dimensione di impresa e dei suoi lavoratori: gli ammortizzatori in deroga sono intervenuti lì. Dovremmo allargare strutturalmente la protezione anche a questi lavoratori, mantenendo la logica della base assicurativa, obbligatoria od organizzata facoltativamente da organismi bilaterali, la cui sperimentazione è in atto e ha dato, tra l'altro, risultati positivi. positivi. Fornirò un quadro dettagliato al Senato della Repubblica circa anche un impiego che è stato gestito soprattutto dalle Regioni, perché le microimprese sono state, in particolare, considerate dalle Regioni per le esigenze di ammortizzatori sociali che hanno manifestato. Così come vorrò dare un quadro riferito all'esperienza degli enti bilaterali, che nell'artigianato hanno concorso ad integrare il reddito dei lavoratori delle imprese associate allo stesso ente bilaterale, che richiedevano una protezione tale da non interrompere il rapporto di lavoro. insomma, continueranno ad essere usati - lo garantisco - anche per il prossimo anno, perché ragionevolmente abbiamo ancora bisogno di strumentazione straordinaria. Allo stesso tempo, presenteremo nei prossimi giorni il piano triennale per il lavoro, nell'ambito del quale verrà descritta soprattutto la riforma che viene chiamata comunemente "Statuto dei lavori", al cui interno ci saranno anche ulteriori disposizioni relative agli ammortizzatori sociali, che si combineranno con l'uso di quella delega prodotta dal Governo Prodi, che il Governo in carica ha accettato, ancorché non dotata finanziariamente.

proprio nel momento in cui abbiamo ricordato lo Statuto dei lavoratori, affermare la centralità della trazione contrattuale nel governo della crisi lungo il vettore della coesione sociale, sia un tema che il Ministro ha colto con grande limpidezza e per questo lo ringrazio.

la richiesta era quella di dare attuazione alla delega, che è stata ulteriormente dilazionata, e di costruire un sistema di protezione realmente universale. degli strumenti modificati in via amministrativa, a noi risulta - e sono dati INPS, che meritoriamente ad aprile ha cominciato a distinguere i dati della Cassa in deroga da quelli più generali della Cassa integrazione straordinaria

che hanno una presenza di piccole e piccolissime imprese molto elevata. Non solo. Questi strumenti avrebbero dovuto tutelare, in larghissima parte, la quota dei lavoratori non garantiti da nessun altro strumento di protezione, i cosiddetti lavoratori atipici

che una riforma realmente universalistica sia indispensabile, perché la crisi perdurerà e, giusto l'altro giorno, il rapporto INPS ci ha detto che gli esuberi nelle imprese aumenteranno.

piccole e medie imprese. Si è iniziato a fare un piccolo passo, ma questa categoria non va abbandonata perché i nostri lavoratori hanno bisogno di sapere che questo Governo continuerà a lavorare per migliorare la situazione.

che non si possono mettere a carico dello Stato ingenti risorse per affrontare le tematiche di cui stiamo parlando questo pomeriggio. Le vorrei allora chiedere semplicemente, se possibile: un'ingente quantità di risorse allo Stato si è potuta chiedere per ripianare il gettito dell'ICI tolta agli abbienti per le loro case, facoltose o meno,

in situazioni drammatiche il Governo ha la responsabilità di dare delle risposte che non siano soltanto di emergenza, ma anche di prospettiva. La domanda mirava a conoscere quali politiche attive, unitamente a quelle passive, e quali risorse il Governo intende mettere in campo per

sia per i lavoratori all'inizio della loro stagione lavorativa che per quelli che devono essere riconvertiti ad altri lavori. Non è questa la risposta che aspettavamo; non sono queste le risposte che possiamo dare né alle parti sociali né ai lavoratori che le aspettano. il Ministro per la sua risposta, ma non ne siamo soddisfatti. L'attuale situazione economica richiede ben altri e decisivi interventi a tutela dei lavoratori da parte del Governo. A nostro avviso, è prioritario che all'uso fin fin qui abnorme dello strumento della Cassa integrazione straordinaria si sostituisca la misura ben più efficace del raddoppio della durata della Cassa integrazione ordinaria: cioè da 52 a 104 settimane. integrazione straordinaria presuppone processi di ristrutturazione e finisce per diventare, di fatto, uno strumento di gestione degli esuberi, mentre la Cassa integrazione ordinaria permette al lavoratore di mantenere il normale rapporto di lavoro e all'azienda di superare la fase di crisi, non perdendo importanti professionalità e competenze, frutto di collaborazioni ed investimenti di anni. Non mi sembra che questo sia la direzione in cui sta andando il Governo, che si appresta, con la prossima manovra, a colpire ancora una volta